Colleghi senatori, Colleghi senatori, vi prego di non iniziare così una seduta che prevede votazioni ed è delicata. Ricordando che vi sono diversi spazi in Senato per

apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, la Presidenza ha ricevuto una pluralità di richiesta di intervento sull'ordine del giorno, a norma dell'articolo 92 Poiché si tratta di una pluralità di richieste su fatti ed episodi diversi, la Presidenza comunica che esse saranno autorizzate a fine seduta, considerata anche l'urgenza di approvare il decreto-legge in scadenza che abbiamo al nostro

16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,

Signora Presidente, come è emerso ieri nel corso della discussione generale, in particolare dagli interventi del relatore e del senatore Pastore, è la terza volta che la legislatura si apre con un decreto-legge che interviene sulla struttura e l'organizzazione del Governo e dei Ministeri. È però la prima volta che questo decreto-legge non aumenta o istituisce nuovi Ministeri, ma attua

questo provvedimento, perché quella legge, che d'altra parte non poteva entrare nel merito, prevedeva semplicemente il richiamo al numero dei 12 Ministeri previsti dalla riforma Bassanini, ma non la suddivisione delle competenze. Con il decreto-legge in esame, quindi, il Governo ha inteso semplicemente limitarsi ad una riorganizzazione sistematica della riforma Bassanini, adeguandola a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008.

autorevoli colleghi verso l'istituzione di un nuovo Dicastero della salute ma, ripeto, questo è semplicemente un decreto-legge di adeguamento a quanto già stabilito dal Senato e dalla Camera con la legge finanziaria 2008 e non pare corretto che in questa sede venga prevista subito una deroga a quelle disposizioni di legge. Noi crediamo che sarà piuttosto l'esperienza di Governo a mostrare, già nelle prossime settimane e nei prossimi mesi,

deroga alla composizione complessiva del Governo, è vero, senatore, che quasi contestualmente con l'emanazione di questo decreto-legge è stata già prevista una deroga, ma, come lei stesso ricordava, essa ha caratteristiche del tutto eccezionali,

stato attuale, il Governo non è intenzionato a prevedere nuove deroghe alle disposizioni previste dalla legge finanziaria 2008. Naturalmente anche in questo caso, senatore Vitali, sarà l'esperienza di Governo e del funzionamento dei buoni rapporti parlamentari a dimostrare se quel numero, fissato dalla legge finanziaria in 60, sia adeguato o no all'efficacia dei rapporti che il Governo intende avere con entrambi i rami del Parlamento e con tutte le Commissioni permanenti. Sicuramente in questa sede vi è la volontà di rispettare, fatta salva l'eccezione che abbiamo richiamato, il dispositivo della legge finanziaria. Sono state poi toccate altre due questioni, sulle quali il Governo brevemente si sofferma adesso

riguardo, per lo spirito del provvedimento, che è semplicemente quello di adeguamento alla riforma voluta dal Parlamento sul numero e la composizione dei Ministeri, il Governo preferirebbe non dare spazio in questa sede a polemiche sull'attribuzione di particolari competenze a un Ministero

senatore Bianco, che ringrazio per la particolare attenzione e competenza, ha rilevato che con il presente decreto‑legge si interviene per un aspetto limitato sulla recente riforma dei Servizi di sicurezza e informazione, che è stata, tra l'altro, voluta nella scorsa legislatura da tutte le forze politiche del Parlamento. È vero che vi è una piccola novella a quella riforma, la quale - come il senatore Bianco sa - è stata introdotta per due esigenze. In primo

secondo luogo, il Governo ha ritenuto, nell'affidare successivamente la delega ad una figura particolare, quale il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio medesimo, di voler rispettare lo spirito e la sostanza di quella riforma dei Servizi. Di fatto l'esclusività è praticamente mantenuta per la figura particolare alla quale la delega

il Senato potrebbe agevolmente procedere a ritirare gli emendamenti che sono stati presentati - il cui spirito il Governo rispetta e in gran parte condivide - e rimettersi all'esperienza dei prossimi mesi di attività

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, ad eccezione che sul comma 22 dell'articolo 1, sul quale il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che siano inserite infine le seguenti parole: del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". In ordine agli emendamenti esprime parere non ostativo ad eccezione che sulla proposta 1.3, sulla quale il parere è di semplice contrarietà, nonché sulla proposta 1.0.1, sulla quale il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, al comma 4, siano inserite in fine le seguenti parole: "Ai componenti del CIPU e del Comitato tecnico permanente non viene corrisposto alcun compenso né indennità né rimborso spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e del Comitato tecnico permanente sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri"». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.100, 1.101, 1.0.1 (testo 2) e 1.500, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

disporre di un Ministero della salute. Il nostro Paese poggia essenzialmente - e sono sicuro che tutti ne convengono - su un sistema sanitario pubblico, che deve basarsi

Signora Presidente, onorevoli senatori, ho ritenuto di presentare l'emendamento 1.2 per recuperare il contenuto

Fu questione già affrontata nelle precedenti legislature e risolta nel senso di porre in capo al Ministero delle politiche agricole e alimentari la prima, immediata fase (non tutta evidentemente) della trasformazione dei prodotti dell'agricoltura.

mi sembra rispondente a logica. Ciò nondimeno, siccome si tratta di una di quelle norme che devono essere armonizzate secondo valenze e criteri sui quali vi possono essere anche punti di vista non ideologici di carattere diverso, auspico che il Governo, nella sua collegialità,

con una motivazione precisa: intendeva restaurare il significato pieno del comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. senza ambiguità escludeva, per il Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità di delegare le sue funzioni in materia ad un Ministro titolare di un Dicastero oppure ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario titolare anche di altre deleghe. consisteva nel divieto all'Autorità delegata dell'esercizio di funzioni di Governo ulteriori rispetto a quelle oggetto della delega.

rafforzare la funzione di *intelligence* e prevedeva, nel contempo, alcuni fondamentali contrappesi, tra i quali - appunto - un limite per il Ministro o il Sottosegretario delegato. Non si trattava quindi di una questione puramente formale. Quella scelta, tra l'altro, fu compiuta fu compiuta consapevolmente, indipendentemente dalla composizione numerica della squadra di Governo. Nel corso del brevissimo esame della Commissione affari costituzionali del Senato è emersa da parte di tutta l'opposizione una sorta di perplessità rispetto a questo comma. sentiti i pareri dei colleghi dell'opposizione, per ragioni per così dire di opportunità occasionale, il Gruppo Italia dei Valori ritira la proposta tendente a sopprimere il comma 21 dell'articolo 1

Onorevoli colleghi, come è giusto che sia, l'opinione pubblica e la stampa, come avrete visto anche questa mattina, seguono con grande interesse e curiosità i lavori delle istituzioni Camera e Senato all'avvio della legislatura. La Presidenza vorrebbe contare sulla collaborazione dei senatori per realizzare un'atmosfera d'Aula e ottenere un livello di decibel compatibili con la comprensione e il reciproco ascolto.

Segnalo altresì che nelle trasmissioni radiofoniche per gli ascoltatori è particolarmente disagevole seguire i lavori del Senato. Mi piacerebbe non dover più intervenire su questo tema,

Abbiamo già spiegato che il fatto che l'Autorità delegata non possa esercitare funzioni di Governo ulteriori finisce per impedire che il Sottosegretario o il Vice Ministro

potrebbe costringere ad un aumento dei Vice Ministri o dei Sottosegretari. Riteniamo pertanto che nell'ambito di tale scelta sia del tutto congruo e logico

Parlamento*. Presidente, al Governo sembrava di aver compreso che il senatore Belisario avesse già accolto l'invito al ritiro.

Si tratta di magistrati che vengono applicati alle dipendenze di un Ministro o di un diverso diverso membro del Governo. Oggi tale applicazione viene stabilita nell'ambito dei diversi

invece che la scelta di questi collaboratori, concordata con i Ministri, avvenga mediante provvedimenti

bene. Infatti, il relatore ha affermato che l'autorizzazione all'applicazione del magistrato avverrebbe con un provvedimento autonomo

come è stato assicurato. Poiché risulta che obiezioni ci sono, la Presidenza non ritiene di poter ammettere l'emendamento Vorrei, inoltre, che le informazioni che pervengono alla Presidenza fossero più puntuali e la Presidenza avesse meglio conoscenza dei rapporti tra i vari Gruppi.

Presidente, prendiamo atto della sua decisione, che d'altra parte interpreta correttamente il Regolamento. una maggiore ed una migliore comunicazione, se vogliamo salvare il *fair play* all'interno di quest'Aula. Non è possibile, infatti, dare informazioni che poi cambiano in corso d'opera; ciò crea un disturbo all'andamento dei lavori che francamente vorremmo evitare, perché altrimenti ci comporteremo di conseguenza.

(testo 2). Infatti, si parla di un Comitato interministeriale per le politiche urbane: il contesto è estremamente interessante, ma una norma di questo genere non si inserisce nel decreto-legge in esame, che riguarda esclusivamente i

La proposta di istituire a palazzo Chigi questo coordinamento interministeriale sui centri urbani è sicuramente interessante ma non riguarda lo spirito del decreto-legge, che è semplicemente di attuazione della riforma sulla composizione del Governo prevista dalla legge

Tra l'altro lei, signora Presidente, proprio in qualità di Ministro, ricorda bene come il Comitato interministeriale per le politiche comunitarie sia strumento utilissimo, che ha dimostrato di funzionare perfettamente: esattamente a quell'esempio

la Commissione bilancio aveva proposto un emendamento, da me accettato, in cui si chiariva che ai componenti del comitato (anche di quello tecnico) non viene corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso spese.

ieri, come ho fatto anche in Commissione, che in sostituzione di questo emendamento avrei presentato un ordine del giorno per impegnare il Governo a non superare

compreso il limite al numero dei componenti il Governo. Noi saremo risolutamente contrari a qualunque ampliamento ulteriore di questo numero; d'altra parte, abbiamo ascoltato anche del rappresentante del Governo che considero importanti, allorquando ha detto che intende rispettare il disposto della finanziaria 2008

parte del relatore e del Governo. «impegna il Governo a verificare la formula normativa più appropriata per risolvere positivamente ogni dubbio

Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la conversione del decreto-legge con cui si provvede al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri non può che incontrare la valutazione positiva del Gruppo Italia dei Valori, dal momento che esso costituisce la prima fase di attuazione di quanto già previsto dall'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), la quale, rideterminando il numero dei Ministeri con rinvio alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo originariamente pubblicato, ha voluto dare un segnale concreto della volontà della politica di varare norme effettive sul contenimento dei costi. L'auspicio è che, nella loro autonomia, tutti i livelli di Governo si adeguino ad un primo esempio di snellimento delle strutture. Altrettanto positiva è la valutazione sulla riduzione dell'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione nelle strutture interessate dal riordino. Il decreto legislativo n. 300, che prevedeva 12 Ministeri, non ha mai avuto applicazione nella sua formulazione originaria. É bene dunque che adesso si torni, seppure con quasi dieci anni di ritardo. Tuttavia, proprio chi come il nostro Gruppo ha sempre sostenuto la necessità di interventi di questo genere ha pieno titolo per ricordare che occorre la massima attenzione, al fine di evitare che la soppressione di alcuni Ministeri ed il riordino che il decreto comporta con il conseguente trasferimento di funzioni, competenze e risorse, determini problemi all'efficacia ed effettività dell'azione di Governo, con conseguenti effetti negativi sull'ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche. La questione riveste importanza sotto un duplice profilo: il decreto in esame comporta una serie di adempimenti successivi che debbono assolutamente porsi come obiettivo di contenimento della spesa e l'ottimale organizzazione interna dei Ministeri oggetto di riordino. Tale fase non sarà semplice, dal momento che già solo la tecnica normativa utilizzata per scrivere il decreto-legge non rende certo trasparente e conoscibile l'effetto, sulle strutture soggette a modifica, delle disposizioni in esame, di non facile lettura e coordinamento. D'altra parte, occorre vigilare anche al fine di prevenire situazioni nelle quali, magari a partire da esigenze meritevoli di attenzione, qualcuno colga l'occasione per ampliare a dismisura il numero dei Ministeri o dei Sottosegretari, ferma restando la necessità per qualsiasi Governo di darsi una struttura capace di interloquire positivamente con le Camere. Ciò non toglie che il nostro Gruppo non tenga nella massima considerazione talune problematiche sollevate nel corso dell'*iter* del decreto-legge in oggetto, a cominciare da quelle concernenti le preoccupazioni per alcuni effetti dell'accorpamento del Ministero della salute nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Abbiamo segnalato nelle Commissioni di merito come ciò possa risultare assai problematico e come riteniamo importante assicurare in ogni caso un coordinamento centrale ed una figura di riferimento autorevole per i problemi del settore sanità, cruciale per l'equità e per la sicurezza sociale. Quale che sia la soluzione che verrà individuata, occorre assicurare il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione e l'interesse della collettività, anche nella prospettiva dell'introduzione del federalismo fiscale,

di quali accorpamenti operare, la scelta di unificare il Ministero della salute e del lavoro, piuttosto che altri Ministeri è stata operata autonomamente dal Governo Berlusconi. Questa scelta, almeno per l'abolizione del Ministero della salute, ha suscitato e suscita molte perplessità. Con riferimento all'ordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, va ricordato come Italia dei Valori avesse espresso, a suo tempo, più di una riserva sul cosiddetto "spacchettamento" dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti operato nel 2006. Se, in linea generale, valutiamo corretto un ritorno all'articolo 55 del decreto-legislativo n. 300 del 1999, che disponeva la nascita del Ministero unificato, riteniamo doveroso chiedere al Governo di salvaguardare il positivo processo di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese di funzionamento e l'opera di riorganizzazione che ha conosciuto il Ministero delle infrastrutture nei due anni appena trascorsi. Si tratta di un lavoro importante che ha iniziato a dare i propri frutti e che sarebbe illogico interrompere. La sua logica va invece estesa, se possibile, alle strutture che tornano, dai trasporti alle infrastrutture. Avevamo inoltre rilevato la presenza di due ulteriori norme che apparentemente non risultavano direttamente riconducibili all'applicazione dei due commi della legge finanziaria per il 2008, a cui il decreto-legge in oggetto si riferisce, ed in particolare l'articolo 1, comma 21, con cui si abroga una parte dell'articolo 3 della recentissima legge di riforma dei Servizi segreti nonché un ulteriore intervento, in sé anche condivisibile, sull'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217. Vista la delicatezza del tema, abbiamo chiesto in Commissione quale fosse la ragione della modifica e quale anche lo stato delle deleghe ad oggi conferite al Sottosegretario in questione (se oltre alle funzioni di segreteria del Consiglio dei ministri, egli abbia una delega semplice per i servizi o sia già «Autorità delegata», del Presidente del Consiglio dei ministri) pronti a valutare con attenzione e rispetto le ragioni sottese all'intervento legislativo. Quello che ci preme sottolineare è come sia interesse di tutti che la confusione sulle deleghe per i Servizi del Presidente del Consiglio dei ministri non arrechi inutili problemi All'Autorità delegata ostacolando l'efficacia delle funzioni di coordinamento e controllo, che sono preziose e non sostituibili nei rapporti col Parlamento.

destra e sinistra votarono l'emendamento relativo a queste norme della finanziaria.Nel momento in cui si parlava di eccessivi costi della politica era inevitabile dare al Paese un minimo di risposta, e questo è stato un ottimo segnale. Oggi, dando attuazione a quella normativa ci poniamo in una

mettendo mano a quelle dinamiche dei costi che sembravano addirittura incomprimibili. Siamo altrettanto soddisfatti che all'interno delle strutture ministeriali dovranno poi essere adottati Regolamenti di organizzazione per contenere le spese. Pertanto, come Lega Nord non possiamo che vedere con favore questo corso della politica, anche se ricordiamo con una certa nostalgia che, per ragioni di contrapposizione politica, una parte di questo Parlamento stimolò il Paese a respingere quella riforma costituzionale che nel 2006 fu sottoposta a *referendum* e che veramente avrebbe un radicale mutamento delle posizioni, dei costi e della specializzazione delle due Camere con la riduzione dei parlamentari. Sarebbe stato quello il momento di dare il segnale al Paese che i parlamentari sanno anche rinunciare

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, proferirò solo poche parole per annunciare il voto favorevole dei senatori del Partito Democratico

del Governo Prodi, a larga maggioranza, da parte sostanzialmente dell'intero Parlamento. Si voleva dare un segnale importante, quello di ridurre drasticamente il numero dei Ministri e dei Sottosegretari ed il decreto-legge va nella direzione da noi auspicata. Sono state introdotte pochissime modifiche, rispetto ad una delle quali avevamo avanzato dubbi e perplessità; mi riferisco, in particolare, alla norma che prevedeva di attribuire l'incarico di Sottosegretario delegato ai Servizi di informazione e sicurezza non, come nella legge di riforma dei Servizi, ad un componente del Governo che si occupasse solo della questione, ma ad un Ministro o Sottosegretario che potesse avere anche altra funzione.

non tanto quella della riduzione del numero dei Ministri e dei Sottosegretari, quanto il fatto che il Governo ha intenzione di affidare tale responsabilità al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che ha la delega anche di Segretario del Consiglio dei ministri, persona che gode di rispetto e considerazione e che ha già svolto con particolare capacità questo incarico nella legislatura 2001-2006, naturalmente ci convincono, ragione per la quale non abbiamo insistito sull'argomento. Le altre questioni sono relativamente marginali. Mi consenta soltanto,

Nelle nostre grandi città infatti si gioca una partita importante per la qualità della vita e per la democrazia del nostro Paese e, naturalmente senza prevedere aggravio di costi, è opportuno che ci sia un migliore coordinamento. Per le ragioni dette i senatori del Partito Democratico voteranno a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.

un *excursus* storico della struttura del Governo. Molti hanno sottolineato che siamo di fronte ad un provvedimento che è esecutivo di norme introdotte nell'ultima finanziaria e che comunque richiamavano la struttura del Governo che derivava

della struttura che tale decreto introduce nell'organizzazione del Governo, una necessità sentita da tutti, soprattutto visto il modo con cui la delega sulla sanità viene gestita dalle Regioni. Ma allora i costi della politica sono riferiti alla funzionalità di talune emergenze che il Paese deve affrontare o ad una struttura che deve costare di meno, al di là della propria funzionalità? Credo che dobbiamo soffermarci su questo dato, perché non credo che il Parlamento

da questo punto di vista messe in condizioni di aumentare i propri costi di gestione dalla sventurata riforma costituzionale che il centrosinistra volle nel 2001. Oggi siamo di fronte ad un sistema delle autonomie locali e delle Regioni che fa lievitare i costi della politica, ad esempio, con l'aumento

rispetto al modello organizzativo del Governo perché dobbiamo dare risposta al dibattito del Paese sui costi della politica. Credo che la democrazia e l'efficienza dell'azione di Governo si debba difendere dimostrando che il Governo che nasce, che ha accettato l'impostazione dell'ultima finanziaria in merito ai numeri e all'organizzazione dell'Esecutivo, ha la capacità di rispondere alle necessità del Paese, modernizzandolo e quindi facendo quelle riforme utili per rispondere alle esigenze di funzionalità della democrazia,

nel tardo pomeriggio di ieri si sarebbe verificato un incidente alla centrale nucleare di Krsko nella vicina Repubblica di Slovenia. Voglio ricordare che questa centrale è situata ad una distanza di circa 100 chilometri dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ed in particolare dalla città di Trieste. Trieste. Ritengo doveroso, quindi, chiedere alla Presidenza un intervento immediato affinché il Governo possa riferire al più presto per comunicare le notizie in suo possesso con riferimento alla natura dell'incidente, alla sua entità

*(PdL)*. Signora Presidente, abbiamo letto sui giornali e abbiamo ascoltato con grande sconcerto dalla televisione che il Presidente della Repubblica, intervenendo in una manifestazione ufficiale ieri a Napoli, ha affermato con grande certezza che i rifiuti tossici portati in Campania provengono dal Nord-Italia. Come italiana mi sento offesa per l'inciviltà del gesto, come meridionale mi sento doppiamente offesa per il fatto che si ritenga che il Mezzogiorno d'Italia debba essere la pattumiera del Nord. Siccome non è stata una frase da comizio, detta da qualcuno di noi come espressione di parte, ma è stata un'affermazione certa e determinata, fatta dal nostro Presidente della Repubblica, ritengo che il Governo debba venire in Aula per relazionare su questo discorso che è estremamente rilevante, anche perché abbiamo avuto Commissioni antimafia e tanti senatori e deputati che sono andati ufficialmente sul nostro territorio per verificare situazioni del genere non vorrei che il denaro degli italiani fosse stato speso per le varie Commissioni ma non per venire a capo di una situazione che definire spiacevole è veramente un eufemismo.

che il Nord debba essere identificato come criminale o che compie azioni illegali nei confronti di un'altra parte del Paese. La magistratura sta svolgendo le sue indagini